Comunico che, in data 30 aprile 2010, e` stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per i beni e le attivita` culturali: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita` culturali»

a conclusione della lettura del calendario, la seduta dell’Assemblea saratolta per consentire i lavori delle Commissioni permanenti, con particolare riguardo al disegno di legge di riforma del codice della strada. L’esame di quest’ultimo provvedimento iniziera domani mattina, alle ore 10, se vi sono le condizioni, previo trasferimento alla sede redigente. Diversamente, saraavviata la discussione generale e il termine per la presentazione degli emendamenti si intende fissato fin d’ora per le ore 19 di domani. Previ accordi intercorsi informalmente tra i Gruppi, la Presidenza potra procedere all’armonizzazione dei tempi. Il calendario della settimana corrente, che prevede anche l’esame di ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri e il seguito del disegno di legge di riforma della professione forense, potrapoi essere integrato con un’eventuale deliberazione – ai sensi dell’articolo 136, comma 2, del Regolamento – sul disegno di legge collegato in materia di lavoro pubblico e privato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e gia approvato dalla Camera dei deputati. La prossima settimana eprevisto l’eventuale seguito del disegno di legge di riforma del codice della strada, nonche´ dei disegni di legge concernenti la riforma della professione forense. Il calendario potra inoltre essere integrato con l’esame del collegato sul lavoro pubblico e privato e della legge comunitaria 2009, ove conclusi dalle Commissioni.